con particolare riguardo all'alluvione di Messina e la situazione occupazionale con particolare riguardo all'attivazione della cassa integrazione guadagni e allo stato di crisi delle imprese, di crisi delle imprese, cui risponderà il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito. Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI. Passiamo dunque alle interrogazioni sul lavoro notturno del personale femminile della CAI S.p.A.; i senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per due minuti ciascuno.

del diritto all'esonero dal lavoro notturno per gli assistenti di volo che siano genitori di minori fino a tre anni di età, o genitori affidatari in via esclusiva di minori fino a dodici anni, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo in materia di tutela della maternità e della paternità. Il citato provvedimento non viene applicato al personale di volo della CAI, dal momento che, nel passaggio del personale da Alitalia a CAI, alle lavoratrice e ai lavoratori suddetti suddetti è stata sottoposta una lettera di assunzione, che è stata sottoscritta dai lavoratori (che sottolineano di averla sottoscritta in assenza di alternative, quindi in termini esclusivi e ultimativi), in cui veniva dichiarata la disponibilità ad effettuare la prestazione di lavoro anche su turni notturni, in contraddizione con i disposti normativi che ho appena citato, ma la frase è riportata testualmente nella lettera di assunzione - «nell'assoluto rispetto della legislazione vigente». L'ambiguità contenuta in questa frase ha dato luogo alle conseguenze cui ci siamo trovati di fronte finora, conseguenze sulle quali sia la giurisprudenza, sia il Ministero hanno dato risposte alternative. Per questo motivo poniamo il quesito, ricordando che il Ministero del lavoro si è espresso in data 22 gennaio sostenendo che per il personale delle compagnie di volo dell'aviazione civile deve ritenersi pienamente in vigore la disciplina dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 che, per l'appunto, dispone l'esonero dai turni di lavoro notturno e dai turni che prevedano il pernottamento fuori dalla sede di residenza; mentre il 4 febbraio del 2009 lo stesso Ministero, con altra risposta risposta ad interpello, ha ritenuto che fossero da escludere sulla materia meccanismi di esonero automatico e che il divieto della prestazione di lavoro dovesse essere disposto solo per le lavoratrici e i lavoratori per i quali fossero riscontrati problemi di salute. Ricordo che la questione coinvolge ad oggi circa 130 lavoratrici e lavoratori con figli minori

Signora Presidente, gentile Ministro, onorevoli colleghi senatori, il contratto collettivo per il personale dipendente della CAI S.p.A. - che, ricordo, è stato firmato il 30 ottobre 2008 con tutte le organizzazioni sindacali di categoria - in materia di maternità e di paternità, all'articolo 21, rinvia espressamente alle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e all'articolo 15 della legge n. 53 del 2000. Inoltre la normativa italiana, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CE, modificata dalla direttiva 2007/73/CE, garantisce alle lavoratrici gestanti e puerpere il diritto di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nelle ore non rientranti nella fascia che va dalle ore 24 alle ore 6, e di concordare con il proprio datore di lavoro lo spostamento in altri orari dei turni rientranti in questa fascia. Sembrerebbe però che nelle lettere di assunzione alle lavoratrici e ai lavoratori della CAI S.p.A. sia stato chiesto di firmare per accettazione una clausola che, se effettivamente apposta nel contratto, equivale ad una rinuncia ad avvalersi dei diritti previsti da queste leggi. Pertanto, oltre a chiedere di verificare se questo specifico addebito alla CAI corrisponda al vero, sono qui a chiedere al Governo se, essendo venuto a conoscenza di questa situazione, non ritenga necessario intensificare l'attività ispettiva di vigilanza presso la CAI, al fine di accertare se esistano realmente le condizioni di violazione della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri.

«per quanto concerne il personale di volo delle compagnie aeree deve ritenersi tuttora in vigore la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001»; di seguito, la lettera cita i casi previsti dalla legge. Lo stesso si trova poi per quel che riguarda i genitori separati, per i quali la relativa disciplina è prevista dalla legge n. 54 del 2006. Purtroppo ad oggi, a distanza di 10 mesi da quella lettera, le richieste delle lavoratrici restano disattese. La situazione di queste mamme nasce da due problemi di fondo: da una parte, la stipula di un contratto capestro, contenente una clausola inosservante della legge; dall'altra, un'interpretazione errata - ci auguriamo in buona fede - che ha comportato la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea

Ad oggi, la CAI continua a non riconoscere i benefici di legge ai propri dipendenti, ma, a seguito di pressioni di vario livello, ha concesso l'esonero dal lavoro notturno esclusivamente ai genitori di figli sotto i tre anni ed ai genitori di bambini disabili, ai sensi della legge n. 104 del 1992. Restano esclusi da questa concessione i genitori unici affidatari di figli fino ai dodici anni, e tutti coloro che hanno a carico familiari disabili. Ricordiamo che la mancata applicazione delle norme di legge comporta un impiego del lavoratore su turni che lo allontanano da casa anche per sei giorni consecutivi, privando i figli ed i disabili delle uniche figure di riferimento capaci di accudirli ed assisterli continuativamente.

Mi permetto solo di fare una considerazione molto breve. La presunta privatizzazione dell'Alitalia, che ha prodotto un carico economico per il Paese e per i contribuenti di circa 6 miliardi di euro nel tempo, e che ha previsto procedure in deroga alla libera concorrenza e al mercato libero europeo nella materia del trasporto aereo, può sopportare tutto, ma non può sopportare anche la circostanza che i famosi capitani coraggiosi che si sono accollati questa grande avventura imprenditoriale scarichino

delle lavoratrici CAI. Clausole vessatorie che dovrebbero essere nulle di diritto, ma che in realtà non lo sono perché il Governo in questa fase non interviene con la determinazione con la quale dovrebbe intervenire per imporre a questi signori, che hanno già avuto un grande regalo da parte dello Stato (e quindi dei contribuenti italiani), l'imposizione di regole fondamentali a presidio della tutela della maternità e della famiglia anche per i lavoratori CAI. Questo è il senso della nostra iniziativa parlamentare e dell'atto ispettivo che oggi le rivolgiamo.

vorrei sottoporre al Ministro una questione che, seppur limitata ad un settore, ad una specifica attuazione, rimanda ad un problema che sta a pieno titolo nell'agenda del mercato del lavoro, della sua opportuna flessibilità e delle sue diverse opportunità. vi è quella della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro delle donne. Una questione che non è certamente risolta a livello generale e che continua purtroppo a costituire un pesante ostacolo sulla strada dell'equiparazione non formale tra lavoratori e lavoratrici in chiave di pari opportunità. Una questione che rimanda a riflessioni più ampie sul ruolo delle donne nei processi di crescita, di sviluppo e della preziosa partecipazione delle stesse al mercato del lavoro e alla ripresa economica che sta davanti a noi, come ci auguriamo. Nello specifico mi riferisco alle clausole che regolano i rapporti di lavoro della nuova Alitalia-CAI S.p.A., laddove si tratta della tempistica con la quale la compagnia provvede alla composizione degli equipaggi dei vari voli per le diverse rotte. Questa modalità operativa che, comprendiamo bene, è ascrivibile alle esigenze di mutevoli e rapide combinazioni di equipaggio, dovrebbe poter tener conto dell'attività di sostegno e del difficile ruolo che anche queste lavoratrici devono ricoprire nei tempi di vita al di fuori del lavoro. Non ci sfuggono, e siamo consapevoli e interessati a sostenerli, i grandi sforzi che Alitalia-CAI S.p.A. sta facendo per recuperare quote di mercato, salvando il destino della nostra compagnia di bandiera e di tanti lavoratori e tante lavoratrici che costituiscono un capitale umano imprescindibile. Le chiedo pertanto, onorevole Ministro, se il Governo non ritenga utile al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla strategia di Lisbona adottare misure ancora più stringenti per le donne, a sostegno della conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli di cura familiare.

gli onorevoli senatori interroganti che consentono al Governo di fornire alcuni elementi di chiarezza - che mi auguro possano essere soddisfacenti - su un tema di grande sensibilità e delicatezza sociale. La materia, come è a conoscenza degli onorevoli senatori, è complessa, necessita di alcuni chiarimenti normativi e investe diversi aspetti. Farò riferimento in primo luogo, come è stato d'altra parte richiamato anche dalla senatrice Ghedini, all'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che configura un divieto generale di adibire al lavoro notturno le donne dal momento della gravidanza fino ad un anno di età del bambino, senza accordare rilievo al consenso di queste ultime, ovvero ovvero ad una diversa volontà, vale dire quella di prestare lavoro notturno. In questo decreto legislativo, come è noto agli onorevoli senatori, è stato individuato un possibile risvolto discriminatorio dalla Commissione europea,

la Commissione europea ha ritenuto che l'automatismo configuri un eccesso di tutela, potenzialmente sfavorevole anche per gli effetti che esso ha in termini di riduzione della retribuzione che ne deriva per la forza lavoro femminile. Tale questione di carattere generale assume poi un ulteriore connotato più specifico per quanto riguarda il personale di volo. Per tale personale, infatti, è controversa l'applicabilità, oltre che del divieto, anche della facoltà di chiedere l'esonero dal lavoro notturno sussistendo le condizioni previste dal già citato articolo 53. Entrambi i profili, quello del divieto e quello della possibilità di chiedere l'esonero, e la posizione della Comunità europea, che aveva individuato un eccesso di tutela sfavorevole nei confronti della forza lavoro femminile, sono disciplinati non solo dal generale articolo 53, ma anche da provvedimenti specifici che trovano invece attuazione per il personale di volo dell'aviazione civile, quali ad esempio il decreto legislativo n. 185 del 2005, citato e che pone una questione di disciplina generale sul lavoro notturno. Il personale di volo che ha problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno o a terra per cui è risultato idoneo. In questo stesso decreto legislativo n. 185 non sono richiamate le disposizioni in tema del divieto di prestare lavoro notturno per la lavoratrice in gravidanza o misure di o misure di tutela in materia di esonero dal lavoro notturno, che sono prese invece in considerazione dal già richiamato articolo 53 del decreto legislativo n.151. Il Governo, in tale complesso quadro normativo, intende attivarsi affinché l'ordinamento italiano sia adeguato alla disciplina comunitaria, modificando l'articolo 53. In particolare, si intende far venir meno il divieto assoluto di lavoro notturno, accordando rilevanza al consenso della lavoratrice, laddove quest'ultima, a fronte dell'accertata non pericolosità per la salute sua e del bambino, ritenga comunque di voler prestare il lavoro notturno. Comunque, va precisato ancora una volta che oggi tale divieto generale non trova attuazione rispetto al personale di volo, a causa di un'espressa richiamata clausola di esclusione contenuta nel decreto legislativo n. 66 del 2003. 2003. Rimane in ogni caso ferma la rilevanza dello stato di salute di ogni lavoratore ed anche della lavoratrice, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 185, rispetto alla questione del lavoro notturno. È prevalente, quindi, lo stato di salute della lavoratrice e, dall'altra parte, il diritto della lavoratrice a chiedere l'esonero rispetto al divieto assoluto, che invece ci è stato contestato dalla Commissione europea. La Commissione europea, infatti (e concludo per questo aspetto della risposta), ha rilevato che la normativa italiana impone un esonero automatico dal lavoro notturno, laddove le direttive europee esonerano le lavoratrici madri dal lavoro notturno solo quando ciò va a detrimento della loro salute e dietro dietro presentazione di relativa documentazione sanitaria. Occorre inoltre considerare la specificità dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile, che è oggetto, com'è evidente, di una disciplina speciale e che considera anche le peculiarità delle attività lavorative e segnatamente il fatto che il pernottamento, anche per periodi relativamente lunghi lontano dal luogo di residenza, rappresenta evidentemente una caratteristica della prestazione lavorativa stessa. Bisogna anche considerare che il già richiamato decreto legislativo n. 185 del 2005 dà rilevanza alle specifiche circostanze che determinano la legittimità dell'esonero dal lavoro notturno per garantire allo stesso tempo un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura dell'attività lavorativa. Si presuppone, quindi, un'articolazione della disciplina della materia che rinvia implicitamente alla contrattazione collettiva per la determinazione delle concrete misure da adottare. Veniamo ora appunto alla materia della contrattazione, che è stata richiamata anche da parte della società CAI.

rinvia espressamente alle disposizioni di legge che sono state richiamate, il decreto legislativo n. 151 del 2001 e l'articolo 15 della legge n. nel contempo delle lettere di assunzione, le lavoratrici e i lavoratori hanno firmato, per accettazione, una clausola - anche qui ricordata - che equivale ad una rinuncia ad avvalersi dei diritti previsti da queste leggi; rinuncia che è ritenuta elemento essenziale del contratto. della rinuncia all'obbligo del divieto di prestare lavoro notturno. Si rileva, infine, che a parte le opinioni diverse in materia, da parte del Governo vi è l'intendimento, comunque, di sostenere ogni iniziativa atta a promuovere una soluzione in via di contrattazione collettiva alle delicate questioni in oggetto, anche per il tramite del ruolo che può essere svolto da parte di tutti gli organi istituzionalmente preposti, incluso l'ufficio della consigliera nazionale di parità. Va ricordato, infatti, che la normativa regolatrice della materia sulla base del principio di specialità è rappresentata dal decreto legislativo n. 185 ed è proprio quest'ultima a rinviare alle parti collettive il compito di individuare la disciplina concreta di tutti i profili qui considerati, incluse le ipotesi specifiche di esonero dal lavoro notturno. Come è stato rilevato anche dalla giurisprudenza più recente che si è occupata della materia, la specificità del settore e, soprattutto, le caratteristiche proprie ed oggettive dell'attività lavorativa prestata, si traducono in rilevanti vincoli di carattere organizzativo in un settore in cui le attività rappresentano un servizio pubblico essenziale. Tutto ciò determina l'impossibilità di poter trasferire in maniera automatica l'impianto complessivo delle tutele che sono offerte dalla legge nella generalità degli altri settori. Rimane dunque la sede della contrattazione collettiva quella maggiormente adeguata a fornire l'idonea regolamentazione della materia, al fine di tener conto per l'appunto di tale specificità ed evidentemente anche dei diritti che sono stati fatti valere in questa sede e rappresentati - credo - in maniera molto efficace da tutti i senatori interroganti.

Signora Presidente, signor Ministro, prendo atto della disamina del problema che lei ha fatto, ma non posso dichiararmi soddisfatta del suo impegno, nonostante ella abbia affermato che la volontà del Governo è quella di portare le parti a trovare una conciliazione. Non posso dichiararmi soddisfatta in relazione agli argomenti da lei richiamati. Innanzitutto, la disciplina europea mette in risalto la volontà delle donne di scegliere se aderire o meno alla prestazione notturna, e qui è assolutamente evidente che proprio in sede negoziale, cioè all'atto della sottoscrizione delle lettere di assunzione, è stata esercitata una coercizione nei confronti di queste donne, che si trovavano in evidente situazione di disparità contrattuale e di potere nei confronti del datore di lavoro; datore di lavoro al quale sono stati riconosciuti da questo Governo ampi margini di discrezionalità e vantaggi imparagonabili a tutte le altre imprese del sistema economico del nostro Paese. È inaccettabile, quindi, che una compagnia che ha un vantaggio competitivo straordinario nei confronti di tutte le altre non riconosca un diritto, che è un diritto soggettivo delle donne - lei stesso lo ha richiamato dicendo competente la consigliera nazionale

ringrazio il signor Ministro. Mi fa piacere sentire che vi è la massima attenzione da parte del Governo rispetto alla problematica evidenziata oggi in Aula. che quest'azione continui con la massima attenzione al fine di evitare che, soprattutto in un periodo di crisi come questo, vi sia la possibilità che qualcuno approfitti della situazione di debolezza dei lavoratori. Auspico, quindi, che l'Esecutivo possa, attraverso un'adeguata attività ispettiva e di vigilanza

di scelta tra il lavoro e la famiglia. Madri e padri costretti a scegliere di rinunciare al posto di lavoro, oppure a far ricorso a tanti congedi parentali o ad altre forme di astensione dal lavoro. Siamo in un caso tipico di Alitalia, rispetto al quale si sta creando un pericoloso precedente; infatti, se il meccanismo dovesse restare impunito, come sta succedendo, altri datori di lavoro senza scrupoli non esiterebbero a far firmare la stessa clausola alle proprie dipendenti

la nostra valutazione è negativa, perché qui non discutiamo dell'adeguamento interno alla normativa comunitaria, del carattere discriminatorio dell'automatismo e quant'altro; queste possono essere tutte argomentazioni condivisibili. Il punto di fondo è un altro: siamo di fronte all'assenza di tutela del contraente debole, la lavoratrice madre, madre, costretta a firmare un nuovo contratto che già prevede un trattamento deteriore sotto il profilo economico e, pur di proseguire il lavoro con CAI, accetta anche clausole nulle e vessatorie come quelle imposte e che lei, Ministro, ha riconosciuto. L'insoddisfazione nasce da una circostanza. Nella vicenda CAI, voi non siete stati terzi, non siete stati soggetti non attivi nella chiusura di un'operazione che costa ai contribuenti italiani 6 miliardi di euro: voi siete stati parte attiva, e non basta dire che vi attivate con la consigliera di parità. Voi dovete chiamare i capitani coraggiosi, questi grandi imprenditori italiani che si sono messi al servizio del Paese

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, apprezzo molto, nella precisione e nella concretezza della sua risposta, l'individuazione dei due temi centrali di questa vicenda. Da una parte, trovo assai interessante e significativo, dal punto di vista dello sviluppo del mercato del lavoro, il ricorso alle alle linee guida europee, che ci invitano a non considerare tutte le garanzie buone per le tutele, poiché tutte le garanzie vanno sempre sottoposte a verifiche, al vaglio del tempo che passa, delle esigenze che si modificano, delle esigenze delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ciò che noi consideriamo una garanzia, talvolta si trasforma in un *boomerang* verso di noi, in particolare nei confronti dei soggetti deboli di questo mercato, e le donne sono ancora indubbiamente uno dei soggetti più fragili del mercato del lavoro. Anche per questo apprezzo il fatto che tutta la *moral suasion* di questo Governo potrà essere utilizzata e spesa perché tra le parti si possa addivenire a una rapidissima soluzione su un aspetto che deve trovare una

signor Ministro, eccezionali eventi alluvionali hanno interessato la regione siciliana negli ultimi mesi e, in particolare, il 1° ottobre scorso la provincia di Messina. I loro effetti hanno coinvolto gli abitati di molte frazioni del Comune di Messina (Giampilieri Superiore e Marina, Molino, Altolia, Briga Superiore e Marina, Pezzolo, Santa Margherita Marina), del Comune di Scaletta Zanclea e del Comune di Itala, determinando la perdita di numerose vite umane e gravi danni ambientali e infrastrutturali. Si chiede di sapere quali iniziative il Governo abbia ritenuto di intraprendere successivamente a favore dei territori colpiti. Altresì si chiede di conoscere le iniziative che il Governo abbia intrapreso per fronteggiare i gravi danni procurati dal violento nubifragio abbattutosi su tutto il territorio siciliano, in particolare nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento, Catania e della stessa Messina, il 16 settembre ultimo scorso, provocando allagamenti, smottamenti, frane, crolli di muri, colate di fango e detriti, esondazioni di corsi d'acqua con il conseguente allagamento di centri urbani e di territori limitrofi, determinando disagi e notevoli danni alla popolazione, alla viabilità, alle linee ferroviarie ed autostradali, agli aeroporti e a numerose attività produttive, nonché interrompendo i collegamenti con alcune isole minori. Per questi episodi la Regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale con le delibere di giunta n. 356/357 del 22 settembre 2009 e n. 408/409 del 30 settembre 2009. Si chiede quindi di sapere quando le delibere siano state trasmesse dalla Regione siciliana al Governo nazionale e quando dallo stesso siano state prese in esame per gli adempimenti successivi di competenza.

in cui noi umani ci siamo organizzati. Invece di far fronte a quei rischi, in questi decenni, abbiamo fatto di tutto per aggravarli e così abbiamo tirato su palazzi, case, persino scuole senza rispettare alcun criterio antisismico; abbiamo cementificato i fiumi costruito laddove non si sarebbe potuto, in maniera abusiva o persino con licenze regolari, abbandonando il territorio senza averne alcuna manutenzione. Il risultato di tutto ciò è drammatico e proprio la tragedia di Messina ce lo ha ricordato nella maniera più luttuosa. Cogliamo l'occasione per esprimere nuovamente il nostro cordoglio ai familiari delle vittime di quella tragedia, che non si può dire né inaspettata né eccezionale.

milioni, una vera e propria elemosina. Si è parlato in questi giorni di un miliardo, che prima doveva essere stanziato dal CIPE e poi doveva essere oggetto di un decreto

per Messina e, più in generale, per questo drammatico problema, o no? Non vi rendete conto che questo è un problema drammatico per la sicurezza dei nostri cittadini? MURA *(LNP)*. Signor Ministro, un'efficace prevenzione del rischio idrogeologico si realizza attuando un'attenta politica di difesa del suolo, attraverso un riassetto del territorio che tenga conto non solo di opere e corsi d'acqua, bensì dell'intera area del bacino idrografico di pertinenza, assumendo la priorità della manutenzione dei corsi d'acqua di montagna, collina e pianura. Anche la salvaguardia delle foreste e in generale la cura dell'ambiente (soprattutto quello montano, con lo sfalcio dei prati e la pulizia del sottobosco) sono interventi in grado di prevenire situazioni di degrado del territorio. Tra le principali azioni per la prevenzione del rischio idrogeologico, risulta fondamentale l'acquisizione delle informazioni di vari fattori di vulnerabilità del territorio e le diverse forme di pericolosità possibili. Qui affrontiamo il discorso del dissesto idrogeologico con particolare riferimento a Messina, ma ricordiamo che questo fenomeno è un denominatore comune in tutto

di cui ben più di 200 sono a rischio frana, più di 400 a rischio alluvione e più di 200 a rischio frana e alluvione. In qualità di parlamentare pavese, non posso fare a meno di citare la tragedia dello scorso 20 aprile, dove, a seguito di precipitazioni atmosferiche incessanti, la collina che sorge sopra la città di Broni, sotto la spinta di fango e acqua, è precipitata. In quel frangente, diverse persone sono rimaste ferite, un'intera palazzina è crollata ed un settantenne è sparito tra le macerie ed è stato ritrovato solo il giorno successivo, ormai deceduto. Pochi giorni dopo, precisamente il 30 aprile, sempre a causa delle abbondanti precipitazioni, è crollato il ponte sul Po di collegamento tra Piacenza e San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. Nel crollo quattro automobili e parecchi passeggeri sono finiti in acqua e, per fortuna, grazie al al pronto intervento della Protezione civile, non ci sono state vittime. Sono questi solo alcuni dei dati che mettono chiaramente in luce la fragilità di un territorio dove bastano ormai pochi semplici temporali, per quanto intensi, a provocare, nel migliore dei casi, allagamenti e disagi per la popolazione. Tale maggiore fragilità è attribuibile ad un uso del territorio e delle acque che troppo spesso non considera le limitazioni imposte da un rigoroso assetto idrogeologico. I primati negativi del rischio idrogeologico nel territorio lombardo sono detenuti dalle province di Sondrio dei comuni è a rischio idrogeologico) e di Bergamo (75 per cento); sempre nella provincia di Bergamo si trova il maggior numero assoluto di comuni a rischio (più di 180). Oltre a tanti piccoli comuni, sono considerati a rischio idrogeologico

Prestigiacomo, visto che questo tipo di rischio ambientale è da considerare una delle maggiori priorità da affrontare per il Paese, per via dell'enorme impatto socio-economico che si determina ogni volta che si verifica un disastro. [LI

da tre settimane era sul tavolo del Consiglio dei ministri uno schema di decreto-legge per la predisposizione di un piano straordinario nazionale contro il rischio idrogeologico da 3-4 miliardi di euro, pensato all'indomani del disastro di Messina e per risolverne l'emergenza. Da quel 3 novembre sono passate altre tre settimane: il il disastro di Messina è del 1° ottobre e sono due mesi che il Governo sta pensando di adottare un provvedimento per risolvere l'emergenza. Inoltre, mentre pensa

passati da 510 milioni di euro del 2008 a 197 del 2009. Insomma, noi vorremmo sapere se il Governo veramente occuparsi della fragilità del nostro territorio. In particolare, vorremmo sapere quali stanziamenti esistano in concreto, con quale finalità e con quale possibile utilizzazione, riguardo al territorio di Messina così devastato dalle alluvioni del 2007 e

nella tragica alluvione che ha visto 38 morti e non si sa più quanti dispersi. Da allora alcune cose sono state fatte, mentre In particolar modo, chiediamo di sapere con esattezza quali siano le risorse a disposizione del Commissario delegato per gli interventi civile, anche considerata la bocciatura di alcuni emendamenti alla finanziaria che servivano a stanziare somme per il rafforzamento delle disponibilità finanziarie necessarie per i primi interventi,

a fronte di uno stanziamento certo che deriva dall'ordinanza della Protezione civile che è pari a 60 milioni di euro. Il Commissario delegato ieri ha annunciato che lo stanziamento non sarebbe di 60

dell'ambiente Prestigiacomo si sarebbe impegnata per uno stanziamento straordinario di 400 milioni di euro a valere sui fondi FAS. Al di là delle chiacchiere e del fatto che solo l'ospitalità negli alberghi per gli sfollati è costata, per per i primi due mesi, oltre 3 milioni di euro e che quindi le risorse stanziate per i primi interventi non sono di per sé sufficienti, non si può continuare così senza avere un quadro chiaro può continuare così senza avere un quadro chiaro di ciò che si vuole fare e di come lo si vuole fare. Vorremmo uno sforzo di verità e di chiarezza, perché credo che lo dobbiamo innanzitutto alle famiglie delle vittime della tragedia dei primi giorni di ottobre che ha colpito la città di Messina e il Comune di Scaletta

all'indomani della tragica alluvione di Messina, stimare in 25 miliardi di euro le risorse necessarie alla riqualificazione ambientale dell'intero territorio nazionale, mentre il Ministro dell'ambiente ha parlato di almeno 3 miliardi di euro per i primi interventi. Si tratta di cifre particolarmente importanti, rispetto alle quali, allo stato attuale, è apprezzabile la decisione del CIPE del 6 novembre scorso di destinare un miliardo di euro a questa materia a valere sulle risorse del FAS. Tuttavia, se consideriamo tutti i tagli che sono stati operati nel comparto in finanziaria, c'è una sorta di contraddizione stridente tra gli annunci alcune decisioni della stessa compagine di Governo. Ci rendiamo conto della mole ingente di risorse che dovrebbero essere messe a disposizione, anche per un periodo di tempo abbastanza lungo, per interventi che dovrebbero rientrare in un piano di salvaguardia nazionale. facendoci carico di questa difficoltà oggettiva, avevamo proposto come Movimento per le Autonomie alcune misure che non avrebbero aggravato il bilancio e avrebbero favorito questo tipo di intervento, ma sono state trascurate e respinte.

con certezza le risorse immediatamente utilizzabili per far fronte all'emergenza e quelle che vengono programmate per gli interventi strutturali di salvaguardia del territorio nazionale,

Presidente, riferirò prima sugli interventi specifici posti in essere dal Governo rispetto agli eventi alluvionali in Sicilia e poi sulle politiche più generali di prevenzione e di tutela rispetto al dissesto idrogeologico sull'intero territorio nazionale, che pure è stato richiamato nelle interrogazioni presentate dagli onorevoli senatori. Per quanto riguarda i vari eventi alluvionali verificatisi il 1° ottobre scorso e che hanno colpito alcuni Comuni siciliani, come noto, il Consiglio dei ministri, in data 2 ottobre 2009, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Messina fino a tutto il 31 ottobre 2010. Successivamente, in data 10 ottobre 2009, è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3815, finalizzata a disciplinare i primi interventi di protezione civile per fronteggiare il contesto critico, porre in sicurezza l'area interessata e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita. A tale scopo, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato con il compito di provvedere in favore dei Comuni interessati al rimborso delle spese sostenute per i primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, alla predisposizione del Piano degli interventi per il ripristino degli edifici e dei beni immobili distrutti o danneggiati ed alla complessiva sistemazione dell'area coinvolta. In particolare, il provvedimento ha autorizzato il Commissario delegato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta o sgomberata un contributo fino ad un massimo di 600 euro mensili, eventualmente integrato da un contributo aggiuntivo, in presenza di altre condizioni di disagio. Per la realizzazione degli interventi fin qui descritti sono stati stanziati 20 milioni di euro a carico delle risorse assegnate alla Regione siciliana nell'ambito dei fondi FAS, 20 milioni a carico del Ministero dell'ambiente ed ulteriori 20 milioni a carico del fondo per la protezione civile nazionale: tutti tali fondi sono stati già trasferiti sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Il Commissario delegato è stato inoltre autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui alla già citata ordinanza, tutte le risorse finanziarie comunque assegnate nonché a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie. Si ricorda inoltre che la rete ferroviaria italiana, oltre ad effettuare i necessari interventi di ripristino delle infrastrutture ferroviarie danneggiate, ha avviato con la Protezione civile regionale una attività di ricognizione sul territorio, volta ad individuare ulteriori situazioni di rischio. Tali necessari interventi saranno inseriti nei programmi gestiti dal Commissario straordinario. È stato dato poi incarico per la realizzazione di uno studio idrogeologico, idraulico e geologico da cui trarre indicazioni per ulteriori interventi migliorativi. Le conclusioni di tale studio saranno portate all'attenzione della Regione siciliana in modo che gli interventi siano programmati in modo concertato con gli altri soggetti interessati. Per quanto riguarda poi un aspetto specifico, oggetto dell'interrogazione del presidente D'Alì, che ha fatto riferimento ad eventi meteorologici avversi che si erano verificati già durante i mesi di settembre e di ottobre e che avevano in particolare investito le Province di Palermo e di Trapani, la Giunta regionale della Regione siciliana, con delibere del 22 e del 30 settembre 2009, ha chiesto al Dipartimento della Protezione civile l'attivazione del procedimento per la dichiarazione dello stato di emergenza. Ma in proposito si evidenzia che tali eventi meteorologici possono in qualche misura essere legati ad altri che hanno interessato l'intero territorio nazionale già nei mesi precedenti e che, come noto, sono stati già oggetto di apposite dichiarazioni di stato dichiarazioni di stato di emergenza. Pertanto, si è ritenuto di predisporre un'apposita disposizione normativa da inserire in una ordinanza della Protezione civile di prossima emanazione, che autorizzi il Presidente della Regione siciliana, già nominato Commissario delegato per il citato intervento calamitoso, ai sensi dell'ordinanza n. 3734 del 2009, a poter utilizzare i mezzi e i poteri straordinari previsti da quella ordinanza anche per fronteggiare il denunciato contesto critico, che in particolare per quanto riguarda le Province di Palermo e di Messina hanno visto verificare dei danni relativi alla sede stradale ed alla sede ferroviaria che hanno riguardato la linea Palermo-Trapani Palermo-Trapani via Castelvetrano, la linea Palermo-Trapani via Milo, e la linea Palermo-Messina, tra Palermo Brancaccio e Bagheria. La circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Trapani via Castelvetrano, in particolare, è rimasta interrotta per oltre 30 ore ed altre interruzioni, sia pure di minore entità, si sono verificate sulla Palermo-Trapani via Milo e sulla Palermo-Messina tra Palermo Brancaccio e Bagheria. L'importo necessario per tali lavori di ripristino, in parte già completati, ammonta a circa 600.000 euro. stati necessari interventi apprezzabili per quanto riguarda i danni che, sempre relativamente ai fenomeni meteorologici del 16 settembre scorso, si sono rilevati all'aeroporto di Palermo, a quello di Trapani e a quello di Pantelleria, che pure in seguito a quegli hanno dovuto registrare ritardi e cancellazioni di voli. Per quanto riguarda la politica più generale del Governo, cercherò di soddisfare le domande degli onorevoli senatori interroganti. Dico innanzitutto che lo Stato ha speso mediamente in questi anni, per la politica di prevenzione dal rischio idrogeologico, circa 350 milioni di euro l'anno

politiche ci sia uno sforzo in tale direzione, che naturalmente il Governo è disponibile ad accogliere. In particolare, i fondi destinati alla difesa del suolo e ad operazioni di prevenzione dal 1991 al 2005 ammontano a circa 5,3 miliardi di euro. Negli anni 2006-2007, per la realizzazione di 644 interventi su tutto il territorio nazionale, sono stati trasferiti agli enti locali ulteriori 416 milioni di euro.

emanare, ricordando solo che nel corso dell'esercizio finanziario 2008 sono stati assegnati alle autorità di bacino di rilievo nazionale altri fondi per circa 16 milioni di euro. Il Governo comunque sta promuovendo il recupero di finanziamenti idonei per intervenire in materia di prevenzione sul rischio idrogeologico. In particolare, l'ultimo CIPE ha recuperato 1 miliardo - com'è stato ricordato - da destinare al programma straordinario per la difesa del suolo; il Ministero dell'ambiente ha aggiunto altri 250 milioni di finanziamento corrente. Inizialmente - è vero - era stato prefigurato un testo di un eventuale decreto-legge, sottoposto all'attenzione del Consiglio dei ministri, al fine di accelerare le procedure di spesa per il dissesto idrogeologico, selezionando le priorità e mediante il ricorso a commissari. Tali indicazioni saranno inserite in un emendamento alla legge finanziaria in corso di discussione alla Camera e per la quale non è ancora scaduto il termine di presentazione degli emendamenti. Conclusivamente, tutti i fondi in questione, sommati ad altrettante risorse regionali, potranno dar vita ad un programma per la difesa del suolo da oltre 2,5 miliardi di euro.

*(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, nella risposta del Governo di oggi si evidenzia l'impegno economico assunto per far fronte alla prima fase emergenziale creatasi a seguito delle alluvioni che hanno colpito il territorio messinese. Non si evidenzia invece un intervento per le alluvioni che hanno colpito il restante territorio siciliano. Da un'attenta analisi non si può che rilevare, però, che tali fondi non sono ancora sufficienti a coprire tutti i gravi danni provocati alle persone e alle cose. Auspico dunque che nella fase successiva il Governo solleciti il Presidente della Regione siciliana, anche nella qualità di Commissario delegato, a definire al più presto l'esatto elenco dei Comuni interessati, della consistenza nel dettaglio dei danni e delle somme necessarie al loro ristoro, anche proponendo l'utilizzo di fondi a disposizione delle intese programmatiche da stipularsi fra Stato e Regione, al fine di ottenere un ulteriore e imprescindibile incremento delle disponibilità nella misura utile a soddisfare le necessità di tutti di tutti i territori colpiti e individuando l'esatta destinazione nell'ambito delle diverse procedure. A me sembra che il confondere alcuni interventi con una procedura nazionale non sia rendere

nella maniera più autorevole possibile, il Commissario delegato ha la disponibilità di quei fondi e li deve spendere. Detto questo, prendo però anche atto che non c'è alcun altro piano straordinario di intervento e mi sembra evidente che rispetto a quanto accaduto a Giampilieri e a Messina quelle risorse risulteranno insufficienti. Più in generale, devo ribadire la mia insoddisfazione perché il ci ha detto che verrà presentato un emendamento. Ora, è vero che non sono ancora scaduti i termini, e vedremo alla Camera che cosa si presenterà, però intanto si continua a procrastinare all'infinito un intervento che, se si voleva fare nella finanziaria, si sarebbe potuto approvare qui in Senato, come già più In particolare, onorevole Ministro, la questione degli stanziamenti per il dissesto idrogeologico non può essere trattata con cifre ballerine, che poi tornano, come i carri armati

vorrei ringraziare il signor Ministro per le risposte che ci ha dato. Mi fa piacere che anche in tale caso, come nel precedente, il Governo abbia dimostrato che c'è attenzione agli aspetti oggi evidenziati

il sottosegretario Menia aveva parlato dello stesso piano, ma mentre il Ministro parlava di un piano da 3-4 miliardi di euro, il Sottosegretario, il 12 novembre, ha parlato di un piano da 254 milioni di euro. Insomma, mi sembra che questa sia un'autentica presa in giro. Avete o no idea no idea di come è ridotto il nostro Paese e della necessità di intervenire con urgenza? semplicemente esterrefatti, e capiamo perché il ministro Prestigiacomo oggi non è qui. Pensavo fosse assente per una delle sue tante gite in giro per l'Italia per fare *reportage* sul dissesto idrogeologico: no, in realtà non è qui perché non sapeva cosa avrebbe dovuto dirci. Fino ad oggi abbiamo ascoltato solo chiacchiere, e siamo al settimo piano straordinario del Governo, dopo quelli antimafia, per le carceri, la sicurezza, la scuola, l'università e le opere pubbliche. L'annuncio di piani straordinari è una presa in giro. Ma la presa in giro in questo caso riguarda le vittime e le famiglie delle vittime di una tragedia di appena due mesi fa.

conforme ad un atteggiamento di responsabilità - che ovviamente non imputo a lei, signor Ministro, che stimo e rispetto per il lavoro che svolge - dire esattamente come stanno le cose e non girare attorno alle chiacchiere e alle promesse quando queste non si possono mantenere. A pagare sono le famiglie messinesi, che in questo momento stanno soffrendo in modo particolare. prendo atto che il Governo ha piena consapevolezza della drammaticità della condizione, sia nello specifico dell'alluvione di Messina sia per quanto riguarda l'intero Paese dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Ma questa consapevolezza non produce ancora

mi fa esprimere un ulteriore rammarico, perché questo ramo del Parlamento non è mai considerato idoneo a compiere scelte importanti, come in questo caso: è sempre una Camera di serie B.

Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la pesante crisi internazionale ha messo a dura prova il nostro sistema economico e industriale. Tale situazione ha fatto emergere come lo Stato sociale italiano sia riuscito a garantire condizioni decorose di vita. In particolare, ciò è stato possibile, tra l'altro, grazie all'impiego degli ammortizzatori sociali e, nello specifico, della cassa integrazione guadagni. Come intende procedere il Governo rispetto all'utilizzo della CIG per i mesi futuri, viste le prossime scadenze della stessa per molte imprese? Sarà possibile, Ministro, proseguire con le attuali deroghe circa la tutela dei lavoratori delle piccole imprese? Infine, vorrei sapere se è allo studio del Governo l'impiego più flessibile della cassa integrazione guadagni, attraverso il conteggio per ore e non per giorni, che comporta una maggiore adattabilità di tale strumento alle diverse esigenze e non, necessariamente, maggiore sfruttamento.

per la CIGS. Ci chiediamo se questi dati siano completi e complessivi e rivolgiamo, quindi, a lei e al Governo questa domanda. Vorremmo soprattutto sapere se il Governo dispone di dati certi sulle casse integrazioni ordinarie in scadenza a fine anno, dato sul quale sia le organizzazioni imprenditoriali che le organizzazioni sindacali stanno lanciando gravi allarmi; se abbia contezza precisa di quanti quanti lavoratori cosiddetti atipici sono stati coperti con gli strumenti in deroga e di quanti, invece, non hanno ricevuto alcuna protezione se, in termini di prospettiva, l'utilizzo degli strumenti in deroga sarà ancora finanziato e se il Governo intende variare il regolamento per l'utilizzo degli strumenti in deroga. È nostra fortissima preoccupazione, infatti, che un utilizzo così ampio (più 700 per cento) degli strumenti in deroga, se ha certamente consentito la protezione di settori produttivi e di lavoratori diversamente esclusi, però configurare una situazione di opportunità impari per i diversi lavoratori e per i diversi comparti che, non avendo pari informazione sulla situazione, non vengono

In Italia il tasso di disoccupazione, da gennaio a settembre 2009, è salito dal 6,8 al 7,4 per cento, ed è assai probabile che tale dato continui a salire nei prossimi mesi, perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico. Nel periodo compreso tra gennaio ed ottobre, sono state richieste 716 milioni di ore di cassa integrazione, un dato quattro volte superiore rispetto a quello del 2008. Ad ottobre il tasso di crescita della cassa integrazione, rispetto all'anno precedente, è stato del 322 per cento per la sola cassa integrazione ordinaria. Per la prima volta in Italia le domande di disoccupazione supereranno nell'anno in corso il numero di un milione. Altissimo è poi il numero dei licenziamenti, drammi che colpiscono migliaia di famiglie, che si ritrovano in pochissimo tempo senza lavoro e senza ammortizzatori sociali. Le chiedo per questo quali iniziative concrete si intendano porre in essere per una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali che porti ad una razionalizzazione dei meccanismi e ad un allargamento della platea dei beneficiari. se non ritenga necessaria l'immediata adozione degli opportuni strumenti normativi volti al raddoppio del periodo di erogazione della cassa integrazione guadagni, e quali iniziative si intendano assumere al fine di evitare il ridimensionamento della presenza

L'altro dato sensibile è la crescita della cassa integrazione straordinaria, e cioè quel sistema che serve a finanziare le crisi strutturali del comparto produttivo e imprenditoriale del nostro Paese. Questo è il dato più inquietante, che si carica di maggior significato se lo leggiamo alla luce delle dichiarazioni che - questa mattina, mi pare - il ministro Tremonti ha fatto in Commissione bilancio alla Camera, dicendo che l'unico deficit che si può produrre in sede di esame della finanziaria alla Camera può riguardare l'eventuale pagamento della cassa integrazione. vuol essere anche il senso della mia domanda - sulla circostanza che manchino i fondi rispetto alla cassa integrazione già autorizzata, e che vi sia una previsione oscura nera sul piano del finanziamento futuro del trattamento di integrazione straordinaria ed ordinaria per i lavoratori, e che quindi la situazione non sia così rosea. Vorremmo sapere con esattezza qual è lo stato dell'arte e delle disponibilità finanziarie in questo settore.

mancando però di sottolineare come si stia registrando anche un'evidente inversione di tendenza, che pare avviarsi definitivamente verso una ripresa economica anche nel nostro Paese. In vista dell'impatto che la crisi avrebbe avuto sul mercato del lavoro, le politiche del Governo sono state mirate, innanzitutto, al potenziamento degli ammortizzatori sociali, anche con riferimento ai lavoratori atipici. Per quanto concerne in particolare gli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione guadagni e mobilità), il Governo ha provveduto stanziando per il 2009-2010 la somma di 8 miliardi di euro. Il Governo è quindi intervenuto a tutela dei lavoratori sospesi o licenziati, potenziando le misure a sostegno del loro reddito con l'indennità di disoccupazione e con l'indennità *una tantum* ai lavoratori co.co.pro.

all'indennità *una tantum* per i lavoratori co.co.pro. per l'anno 2009 è stata destinata la somma di 200 milioni di euro. Infine, è stata prevista un'ulteriore indennità *una tantum* a favore dei lavoratori somministrati, privi di ogni altra forma pubblica di sostegno al reddito, e tale indennità, pari a 1.300 euro, al lordo delle trattenute di legge, ha visto uno stanziamento complessivo di 40 milioni di euro. Per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni straordinaria, relativamente alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa a regime, la legge finanziaria per il 2009 ha previsto lo stanziamento di 600 milioni di euro ai fini delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga. Sugli ammortizzatori sociali in deroga, ricordo inoltre l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, che ha assegnato per gli anni 2009-2010 risorse pari a 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale occupazione e formazione. Questi sono i dati relativi agli interventi del Governo a favore di questi indispensabili strumenti. Naturalmente, era prevedibile che gli effetti della crisi economica, di portata mondiale, alla quale abbiamo assistito nel 2008-2009 portassero ad un massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni da parte del sistema produttivo italiano. È per questa ragione che il Governo era preventivamente intervenuto con i finanziamenti ai quali ho fatto riferimento. Nei primi dieci mesi del 2009, è stato effettivamente registrato un incremento dell'utilizzo di tali strumenti rispetto allo stesso periodo del 2008: in valore assoluto sono state 716 milioni le ore complessivamente autorizzate di cassa integrazione guadagni; però, su base mensile, si registra un'inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti: la cassa integrazione guadagni di ottobre 2009, anche in relazione agli andamenti stagionali degli anni precedenti, sta mostrando una controtendenza. Rispetto al mese di settembre vi è infatti una riduzione delle ore autorizzate pari al 9,7 per cento; in valore assoluto, una riduzione di oltre 10 milioni di ore. L'analisi delle gestioni ottobre 2009 su settembre 2009 fa inoltre rilevare una flessione della cassa integrazione guadagni ordinaria del 17,6 per cento e un contenuto aumento, pari al 5 per cento, di quella straordinaria, dovuto principalmente alla cassa integrazione in deroga. Al momento, quindi, si evidenzia che si sta registrando un minor utilizzo e ricorso alle ore di cassa integrazione ordinaria rispetto alle ore che vengono autorizzate alle aziende. L'ISTAT, nel mese di settembre 2009, ha comunque rilevato un miglioramento degli indici congiunturali e del fatturato degli ordinativi, che nel confronto con il mese precedente hanno registrato, rispettivamente, incrementi del 2,3 e del 5,2 Il fatturato delle imprese è aumentato dello 0,1 sul mercato interno, e del 7,7 su quello estero. Gli ordinativi nazionali hanno registrato una crescita del 4,2 per cento, e quelli esteri del 7 Il PIL, nel terzo trimestre 2009, è aumentato dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente, principalmente nei settori dell'industria e dei servizi. In definitiva, si può quindi affermare che il tessuto produttivo italiano sta reagendo nel modo migliore alla crisi economica, e che sono già diversi i segnali confortanti che fanno intravedere spiragli di possibili miglioramenti nel 2010, anche se, probabilmente ed evidentemente, le conseguenze in termini di occupazione e di mobilità saranno, come sempre è avvenuto anche in passato, proprio le più lente a normalizzarsi. Proprio per questo, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, è stata promossa la definizione di una strategia di interventi per le situazioni di crisi industriale che, attraverso la struttura per le crisi di impresa istituita presso la Direzione generale per la politica industriale e la competitività opererà dando concreta attuazione a tutti gli interventi previsti dalla recente "legge sviluppo". In particolare, e concludo, tale legge prevede la riforma degli interventi di reindustrializzazione attraverso la definizione, sulla base di criteri aggiornati, delle aree di crisi industriali, e la previsione di uno strumento di accordi di programma per l'adozione di interventi, di concerto con il Ministero del lavoro e le Regioni interessate, che permettano di contribuire alla risoluzione delle situazioni complesse. Le risorse per i predetti interventi sono già assicurate dallo stanziamento approvato dal CIPE lo scorso mese di giugno. Ministro, la ringrazio per la risposta, che mi conferma che vi è da parte del Governo un'attenzione verso il tema del lavoro in Italia. Particolare sensibilità è già stata dimostrata in materia di flessibilità, di cassa integrazione guadagni, nel nuovo sistema di conteggio in giorni e non più in settimane, consentendo alle imprese di poter di fatto applicare la cosiddetta settimana corta. Particolare attenzione dovrà comunque sicuramente essere dedicata alla piccola impresa, con la maggior utilizzazione possibile dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga. GHEDINI *(PD)*. Signor Ministro, purtroppo la sua risposta è semplicemente un commento ai dati di cui disponiamo già, e non diminuisce la nostra preoccupazione, anzi la acuisce, la acuisce, perché rimane forte in noi il timore che manchi nel Governo una visione prospettica della crisi, e soprattutto dei modi per uscirne. È stato detto in tutti gli interventi - e lei lo ha ripetuto - che l'utilizzo massiccio e straordinario degli ammortizzatori richiede una loro modifica e una loro riforma. Ancora questa mattina in Aula la stessa affermazione è stata fatta da autorevoli rappresentanti del Governo, che però nel contempo hanno nuovamente dilazionato la riforma a dodici mesi, e oltre, da oggi. Per quel che riguarda gli stati di crisi, la gestione centralizzata dei medesimi e l'impossibilità di accesso uniforme

la ringrazio per la risposta, ma siamo abbastanza pessimisti rispetto all'inversione di tendenza che lei oggi ha voluto segnalarci. Vorrei infatti sottolineare la necessità di intervenire subito su una situazione difficile per tante famiglie; se non ci sarà un intervento tempestivo, diventerà davvero tragica. È necessaria - ripetiamo da tempo - un'articolata riforma degli ammortizzatori sociali: ma subito, non tra due anni, come avete stabilito questa mattina lavoro (disegno di legge n. 1167). È necessario che quelle poche risorse che il Governo ha a disposizione vengano investite, non in opere faraoniche o nel progetto della *social card*, un progetto fallimentare, fallimentare, ma - lo ripetiamo - sul mercato del lavoro, dove la situazione, tra cassaintegrati, precari e disoccupati sta esplodendo: abbiamo visto anche questa mattina tanti che protestano nelle piazze. le previsioni di autorevoli istituti non sono rosee. Si prevedono infatti per fine anno 500.000 disoccupati in più. Tutto ciò metterà le famiglie in ginocchio, per cui vi preghiamo di intervenire davvero concretamente.

di una riduzione del 17,6 per cento del ricorso alla cassa integrazione ordinaria, che è lo strumento che per sua natura viene utilizzato per far fronte alle cosiddette crisi di carattere congiunturale, cassa integrazione straordinaria è uno strumento di sostegno ai lavoratori in caso di crisi aziendale a carattere strutturale. Questo è il dato che cresce e che determina lo scivolamento della crisi verso la sua strutturalità, su cui non vi sono politiche adeguate da parte del Governo. Ciò è confermato dalle dichiarazioni del ministro Tremonti, che annuncia la possibilità di toccare i saldi di bilancio nella legge finanziaria solo per finanziare ulteriori interventi relativi agli ammortizzatori sociali, mentre il resto degli interventi dovrebbe essere finanziato con il gettito dello scudo fiscale. Pertanto restiamo maggiormente preoccupati, perché abbiamo una lettura totalmente diversa di quei dati, e credo che ce l'abbiano tantissimi operatori economici.